fotografa ancora una situazione di crisi, con ombre, che peraltro vengono da lontano, e qualche luce. Il Paese, a causa dei problemi strutturali ormai atavici, fa ancora fatica ad invertire la rotta. La rigorosa politica di bilancio avviata nella scorsa legislatura, in particolare dal Governo Monti, politica che ha imposto sacrifici agli italiani, ma che ci ha permesso anche di uscire dalla procedura di *deficit* eccessivo avviata nel nel 2009 dalla Commissione europea e che dovrebbe farci centrare l'obiettivo di medio termine del pareggio strutturale (auspichiamo però che il prossimo anno, in occasione della Presidenza di turno

Infatti, se analizziamo attentamente gli indici relativi all'esercizio 2012, riscontriamo un parziale miglioramento di alcuni saldi ottenuti proprio grazie alle manovre di correzione dei conti pubblici per il 2012. Nonostante il PIL abbia registrato una flessione del tasso di crescita del 2,4 per cento, l'indebitamento netto è sceso a 47,6 miliardi, pari cioè al 3 per cento del PIL, rispetto al 3,8 per cento registrato alla chiusura dell'esercizio dell'anno scorso, dato che - vale la pena ribadirlo - ha consentito al nostro Paese di uscire dalla procedura di *deficit* eccessivo. L'avanzo primario è risultato positivo, pari al 2,5 per cento, in miglioramento di 1,3 punti percentuali rispetto al 2011. Certo, il debito pubblico ha subito un incremento, raggiungendo la ragguardevole cifra di 1.988,66 miliardi di euro. Va osservato comunque che nell'area euro solo l'Italia e la Germania hanno fatto registrare ampi avanzi primari. Quindi, il 2012 è stato effettivamente un anno molto duro per l'intero Paese. A questi dati dobbiamo poi affiancarne altri che mettono chiaramente in evidenza una realtà socio-economica ancora in forte disagio, come peraltro già denunciato nel DEF che abbiamo avuto modo di esaminare alcuni mesi fa. La domanda interna, infatti, è scesa, il tasso di disoccupazione è salito, i prezzi al consumo, a fronte di un livello delle retribuzioni pressoché invariato, sono saliti del 3,3 per cento, la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici nel primo trimestre 2013 è stata pari al 9,3 per cento (in aumento di 0,9 punti percentuali rispetto al trimestre precedente) e la pressione fiscale si è attestata al 44 per cento del PIL, quasi tre punti superiore alla media degli altri Paesi della zona euro. Quest'ultimo dato, in particolare, ci deve far riflettere sulla necessità, peraltro proprio in questi giorni annunciata dal presidente del Consiglio Letta, di un intervento mirato alla revisione del nostro sistema fiscale per alleggerirne il peso sul lavoro, sull'impresa e sulle famiglie. un'operazione certamente non facile, anche per le significative differenze territoriali che si sono determinate nel tempo per quanto riguarda il prelievo a carico delle famiglie e delle imprese. Mi riferisco in particolare alle addizionali regionali e comunali, di cui oggi parlano anche alcuni quotidiani, le le cui aliquote differiscono molto da Regione a Regione e da Comune a Comune. Auspichiamo quindi al più presto un intervento in questo ambito, proprio per spostare e riequilibrare la pressione fiscale rispetto al lavoro, magari facendola pesare maggiormente sulla cosiddetta rendita. rendita. È una fotografia panoramica quella che del nostro Paese danno i provvedimenti oggi al nostro esame (e mi riferisco al rendiconto). Ma sappiamo tutti benissimo che la fotografia è un'immagine statica, scattata in un momento particolare; ora, però, a quello scatto ne stanno seguendo altri, che offrono immagini nuove e in molti casi anche migliori. Infatti, il Governo e il Parlamento hanno varato una serie di importanti provvedimenti che stanno cambiando e cambieranno significativamente quell'immagine di cui ho parlato. Per citarne solo alcuni, ricordo il decreto che ha sbloccato i pagamenti della pubblica amministrazione e, stando alla nota ricevuta dall'ufficio stampa del Ministero dell'economia e delle finanze, aggiornata al 4 settembre, risulta che siano stati messi a disposizione degli enti pubblici debitori ben 17,9 miliardi di euro, (quasi il 90 per cento dei 20 miliardi stanziati con il decreto-legge n. e che questi abbiano provveduto a pagare i propri debiti scaduti per un importo pari a 7,2 miliardi di euro, cioè il 36 per cento dell'importo stanziato. Rispetto al precedente aggiornamento, che risale all'agosto scorso, il monitoraggio ha fatto registrare in poco tempo un incremento di 2,2 miliardi nei pagamenti effettuati ai creditori. Ci auguriamo ovviamente che il Governo faccia ancora di più per accelerare i pagamenti

Inoltre, come sappiamo, il decreto-legge n. 102 del 2013, emanato dal Governo il 31 agosto scorso, prevede il pagamento di altri 7,2 miliardi di euro dei 10 miliardi aggiuntivi ai 20 già stanziati nel corso del presente anno; questo si tradurrà per le imprese creditrici in maggiori benefici in termini di investimenti, produzione e consumi: in nuovi stimoli per la politica del credito. Per questi motivi, noi del Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, consapevoli del fatto che si tratta di una misura eccezionale per un Paese in forte crisi di liquidità, abbiamo votato a favore dell'emendamento presentato dal Governo in Commissione sul disegno di legge di assestamento del bilancio, volto ad incrementare di ulteriori 18 miliardi l'importo massimo dell'emissione dei titoli pubblici, portandoli a 98 miliardi totali, in quanto riteniamo che tale modifica consentirà, visti i tassi di interesse ancora sostenibili, di garantire il finanziamento del fondo per i debiti della pubblica amministrazione, di poter contare su un maggior gettito IVA di affrontare i primi mesi del 2014 con una sufficiente riserva di liquidità che ci consentirà di avviare i primi passi verso la ripresa economica. il decreto del fare, che abbiamo approvato prima della pausa estiva, i cui effetti reali positivi potremo valutare solo nel prossimo anno, in occasione dell'esame del rendiconto e dell'assestamento del 2013. Così come potremo valutare gli effetti del citato decreto-legge n. 102, che prevede una serie di misure molto attese, come il rifinanziamento della cassa integrazione guadagni, un'ulteriore salvaguardia dei lavoratori dall'innalzamento dei diritti di accesso al pensionamento (cosiddetti esodati), misure a sostegno delle famiglie sui mutui per la prima casa e gli affitti e l'abolizione definitiva della prima rata IMU dovuta per il 2013 per le abitazioni principali, nonché per le aree agricole.

e, soprattutto, che sia ispirata ad una logica federalista che dia la possibilità ai Comuni di gestirla con grande flessibilità, come avveniva, per certi versi, con la vecchia ICI. ICI. Nonostante le recenti proiezioni dell'OCSE che danno l'Italia come unico Paese del G7 ancora in recessione, noi del Gruppo Per le Autonomie siamo fiduciosi. Siamo convinti infatti che il lavoro di questo Governo di necessità e di servizio ci farà agganciare la ripresa che si sta delineando nell'eurozona, una ripresa confermata anche dall'EUROSTAT, che ha certificato per il secondo trimestre una crescita del PIL dello 0,3 per cento rispetto al primo trimestre di questo anno. A questo proposito anche dalle informazioni riportate nella relazione al Parlamento presentata dal Presidente del Consiglio...

Uffici, concludo facendo una considerazione. Oggi come oggi stabilità, certezza, dialogo e collaborazione fra tutte le forze politiche sono gli ingredienti necessari alla buona riuscita o, meglio, all'uscita del Paese: dalla fase non possiamo permetterci di dimenticare e tralasciare solo uno di questi ingredienti perché significherebbe mettere in ginocchio definitivamente il nostro Paese, che non lo meriterebbe. Pertanto il Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE voterà a favore dei due provvedimenti oggi in esame. *(Applausi

che, a nostro avviso, non è adeguata alla situazione economica del Paese: riproducono una visione di austerità, di contenimento eccessivo della spesa, soprattutto di quella che noi dovremmo destinare, così come è stato fatto in altri Paesi del sistema internazionale occidentale, agli investimenti, in particolare a quelli produttivi

non solo questo, ma anche quello precedente - ha presentato in questa fase. È una modalità pressoché esclusivamente burocratica, chiusa nelle stanze di coloro che conoscono perfettamente le procedure di contabilità, ma che non hanno l'animo o, meglio, l'anima necessaria per ascoltare i problemi del Paese. i problemi del Paese. Noi abbiamo stima per le abilità che anche questo Governo contiene; abbiamo stima personale ed anche considerazione nei confronti del Presidente del Consiglio. la stima personale e la considerazione non bastano per condividere un orientamento di maggioranza, una gestione un po' troppo articolata degli orientamenti di politica economica che devono fare i conti con la divaricazione di tipo politico presente sistematicamente espressa platealmente dalle diverse posizioni nella politica economica e in quella fiscale

In questa stessa Aula, non più tardi di qualche mese fa, abbiamo approvato unanimemente un ordine del giorno in cui si invitava il Governo a non consentire l'approvazione dei bilanci preventivi delle amministrazioni locali il 30 settembre, cioè ad anno inoltrato, anzi quasi concluso. La risposta è stata data nell'ultimo decreto emanato dal Governo, che ha spostato la data per l'approvazione dei bilanci preventivi dei Comuni dal 30 settembre al 30 novembre. Io ho suggerito di spostare al 31 gennaio 2014

quelle responsabilità politiche fanno alle loro comunità, ai loro cittadini: raccontano come spenderanno i soldi. Ma come fanno a raccontare come spenderanno i soldi e a dare la possibilità di intervenire

sono sempre più ristretti, sempre più circoscritti a modalità di natura contabile, ad un approccio che - a nostro avviso - è troppo burocratico e non ha anima. Grazie il rendiconto generale e l'assestamento di bilancio sono provvedimenti che solitamente non trovano all'interno della discussione politica il tempo e lo spazio che invece meriterebbero (abbiamo avuto modo di verificare l'andamento dei lavori). È pur vero che la mole di documentazione la complessità dei due provvedimenti potrebbero far desistere anche la persona più curiosa: in Commissione quanti fascicoloni erano stai stampati! È altresì vero, Presidente, che, mentre il rendiconto fotografa perfettamente lo stato dell'arte delle entrate e delle uscite relative all'anno precedente, l'assestamento evidenzia invece gli impegni che il Governo intende assumersi sia per il presente che per il futuro. E questi documenti meritano un'attenta analisi. Non è intenzione mia, né del mio Gruppo, snocciolare tutti i dati contabili; ci pare invece opportuno evidenziare alcuni aspetti importanti.

(ricordo che l'anno scorso il Governo era presieduto dal professor Monti). Il valore del PIL - forse il maggiore degli indicatori economici - è quello che più di

che, sommati al dato negativo del 2012, che oggi vediamo cristallizzato nel rendiconto, rappresentano un macigno sulle già fragili spalle dell'Italia. Una situazione economica così configurata non lascia certamente spazio a proclami di ripresa: anzi, i dati che emergono dai provvedimenti evidenziano piuttosto che le politiche economiche adottate negli ultimi mesi sono state profondamente recessive.

La forte pressione fiscale, congiuntamente all'imposta immobiliare sulle attività imprenditoriali, ha avuto ulteriori effetti depressivi, determinando un vero crollo dei consumi e, conseguentemente, del gettito IVA. Ricordiamo che questo Governo aveva promesso di togliere l'IMU sui fabbricati degli imprenditori perché si tratta di attività che a loro servono per vivere e fare PIL; non ha però mantenuto questa promessa. È evidente che la negativa dinamica economica non favorisce assolutamente una ripresa. È però altrettanto palese che le negative scelte politiche adottate, basate su una forte contrazione della spesa di investimento (guardate bene: investimento, non spesa corrente), hanno ulteriormente concorso ad aggravare una situazione già di per sé drammatica. Tutto questo mentre nel resto dell'Europa i diversi Governi nazionali adottavano scelte di rilancio dell'economica nazionale:

Adesso stanno a meno di noi: questo significa che il Governo spagnolo ha messo in atto politiche economiche per favorire la ripresa economica. Il Governo italiano, ora presieduto dall'onorevole Letta, non ha fatto nulla.

Dati negativi, quindi, su cui il Governo non ha provveduto e continua a non provvedere con concrete azioni di tagli della spesa pubblica. Tutt'altro. I dati evidenziano come i conclamati provvedimenti di taglio della spesa pubblica non hanno ancora dato i frutti sperati: aumenta la spesa corrente, viene ridotta, quasi per compensare tale aumento, la spesa capitale. Un dato, quest'ultimo, assolutamente controproducente: come tutti noi sappiamo, infatti, sono proprio le spese di parte capitale a permettere il rilancio economico del Paese, rappresentando queste le risorse che poi vengono utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche. Di fronte a tutti questi dati è già partita la gara dello scaricabarile per individuare i responsabili di una situazione al limite del baratro, con un Governo Letta che vivacchia quotidianamente, millantando sui *media* provvedimenti risolutivi.

di questa tradizione, si cerca di far credere ai cittadini che si pone rimedio ad un proprio provvedimento, senza considerare che la coperta è sempre più corta, proprio a causa di azioni scellerate e politiche miopi, giustificate dalla necessità di incassare risorse fresche nel breve periodo. mentre i Comuni virtuosi hanno il mal di testa per programmare i propri bilanci, quelli spendaccioni continuano a gettare denaro dalla finestra. I fondi per alcuni Comuni, presenti nel bilancio di assestamento, gridano vendetta, onorevoli colleghi,

piuttosto che la scoperta di interi Paesi abusivi, come quello di Torre Mileto, non fanno altro che avvallare, purtroppo, sempre più la nostra posizione politica, immutata, a differenza di altri Paesi, da vent'anni a questa parte. *(Applausi dal vedere una luce in fondo al tunnel, se davvero vogliamo credere in una ripresa, dobbiamo prima di tutto intervenire sul debito pubblico, eliminando per sempre quelle inefficienze e iniquità che continuano ad affossare il nostro Paese. noi voteremo contro sia al rendiconto che all'assestamento Signora Presidente, colleghe e colleghi, il Gruppo di Scelta Civica voterà a favore di entrambi i disegni di legge si ritrova nelle considerazioni dei relatori e anche nell'intervento del rappresentante del Governo, il sottosegretario Giorgetti. Il mio collega Olivero ha ricordato nell'intervento di ieri che il bilancio gli atti conseguenti sono uno specchio della situazione economica, politica e sociale del Paese. Se così è, questo strumento, come gli strumenti collegati, appunto il rendiconto e l'assestamento,

che pochi in quest'Aula possano comprendere i meandri di volumi e volumi depositati presso la 5a Commissione e che sono, appunto, oggetto della votazione di oggi. Su questi due atti contabili ci sono i segni di un percorso virtuoso di riequilibrio dei conti pubblici, e solo una polemica distruttiva, come è spesso quella italiana, non considera il percorso che abbiamo positivamente compiuto. Su questi due atti contabili ci sono anche i segni dei sacrifici compiuti dagli italiani, da tutti noi, per il riequilibrio di questi conti di questi conti e ci sono anche i segni dell'avvio di una politica di rilancio. Voglio estrapolare alcuni elementi da questi due provvedimenti, senza certamente esaminarli nella loro interezza.

penso, senatrice Comaroli, che non sia affatto un problema del Governo Monti, ma un problema che veniva da lontano, il fatto che il PIL nel nostro Paese da tanto tempo soffriva, calava, non cresceva),1

il saldo primario - come è stato ricordato in quest'Aula - è il migliore, dopo quello della Germania, di tutti i Paesi dell'Unione europea. C'è stata una nuova riduzione dell'indebitamento, superiore a quella che si era registrata in tempi migliori, e anche nella gestione di competenza c'è un saldo netto positivo. Quindi, in quest'Aula si dimentica spesso come ci trovavamo nell'autunno del 2011, contenuti, appunto, nel rendiconto del 2012. Oggi collochiamo il decennale BTP al 4,46 alla fine del 2011 e nel corso di una parte dello stesso anno i decennali erano collocati al 7,50 Va quindi apprezzata l'opera del Governo Monti e oggi va dato atto che il Governo Letta, nonostante i problemi e le turbolenze politiche, riscuote credito. In questo rendiconto c'è anche il segno del grande lavoro e dei sacrifici compiuti per non cadere nel baratro economico-finanziario. E nonostante ciò, a ricordarci che la crisi non è superata affatto, la crisi dei conti pubblici, abbiamo un *rating* preoccupante. In questo rendiconto 2012 ci sono anche i segni dei non pochi provvedimenti intervenuti nel corso del 2012, e anche alla fine del 2011, per produrre effetti di riduzione della spesa pubblica. Una spesa che, non dimentichiamolo mai, sconta anche il nostro apporto significativo ai meccanismi europei di stabilità finanziaria.

grave crisi economico-finanziaria, abbiamo comunque contribuito a cercare di risollevare le sorti economico-finanziarie di altri Paesi dell'Unione europea. E tra le misure di una certa rilevanza ci sono le novità in materia di acquisto di beni e servizi della pubblica amministrazione. Siamo intervenuti, i Governi sono intervenuti, sono intervenuti, sul pubblico impiego attraverso la riduzione del *turnover*, la razionalizzazione della pianta organica e il blocco dei salari e degli stipendi.

il rapporto non virtuoso tra salari e stipendi bloccati da tempo del pubblico impiego e il merito, per aumentare la produttività della pubblica amministrazione. Poi ci sono le manovre varate nel corso del 2011 e del 2012: cito una per tutte, quella dell'aumento dell'IVA dell'1 Sull'assestamento per il 2013, l'altro provvedimento, certo, constatiamo un peggioramento netto del saldo finanziario di bilancio. Questo peggioramento, però, non è doloso, come tante volte è avvenuto in passato frutto di una dissennata politica della spesa (ci ricordava il sottosegretario Giorgetti un andamento in passato poco attento): è principalmente il frutto di scelte politiche che sono state compiute dal Governo Monti e, oggi, dal Governo Letta.

per intervenire con un provvedimento *ad hoc* sui ritardati pagamenti della pubblica amministrazione. L'assestamento registra anche minori entrate finali, che sono effetto di una difficoltà oggettiva nel quadro della crisi economica: la contrazione dei consumi che ci fa incassare meno IVA, e altre imposte, accise e via dicendo. Il tutto è parzialmente bilanciato - molto parzialmente bilanciato da un incremento delle imposte sia sulle persone fisiche che sulle società, probabilmente per una intensificazione della lotta all'evasione e all'elusione.

degli stipendi della nostra gente, del reddito delle nostre persone, del nostro popolo. La medicina è la crescita:

Mentre in Italia infuriano i dibattiti politici e giudiziari, in Europa e nel mondo ci sono segnali che sarebbe un peccato sprecare: basti pensare ai bassi tassi che si mantengono ancora in tutto il mondo economicamente avanzato. Questo è il momento della stabilità, proprio perché abbiamo raggiunto il riequilibrio dei conti pubblici. É il momento di dare corso agli impegni più robusti assunti sulle riforme strutturali, sulla riduzione della spesa pubblica e sugli stimoli alla crescita. il rendiconto rappresenta quello che lo Stato ha fatto in un anno. Appare inconcepibile che fino a questo momento le forze politiche abbiano concentrato tutta la loro attenzione sul bilancio preventivo, disinteressandosi di quanto effettivamente poi accada.

La prassi-sistema che si è sviluppata è quella della cogestione, dove le forze politiche fanno finta di scontrarsi sul bilancio preventivo, ma di fatto decidono insieme sulla grande parte dei provvedimenti. Ora la maggioranza PD e PDL ha messo nero su bianco questa prassi di corresponsabilità. Si dice una cosa, bilancio preventivo, e si fa il suo opposto, bilancio consuntivo. La prima cosa che salta all'occhio è la premessa nel disegno di legge: «In Italia le tensioni registrate sui mercati finanziari nella seconda metà del 2011 hanno indotto una forte irrigidimento delle politiche di bilancio, mirate a centrare l'obiettivo di medio termine del pareggio strutturale e la chiusura della procedura per *deficit* eccessivo aperta nel 2009». Pertanto, gli ultimi tre Governi che si sono succeduti si sono posti l'obiettivo di far quadrare i conti dal lato della spesa, imponendo si fa per dire - a ciascun Ministero la riduzione delle dotazioni finanziarie e prevedendo che fossero le amministrazioni a proporre su quali stanziamenti effettuare riduzioni e, solo qualora ciò non fosse stato fatto, il Ministero dell'economia e delle finanze sarebbe intervenuto con tagli lineari, attuati con gli occhi bendati però. Il risultato è stato che si è tagliato male e alla cieca nel ventre molle degli italiani, riducendo il finanziamento agli enti di ricerca e bloccando gli stipendi pubblici, per nulla rinunciando agli enti inutili, anzi creandone di nuovi, per ultimo la nomina di un ennesimo commissario super esperto che farà una ennesima relazione sulla spesa pubblica, che per l'ennesima volta giacerà in un cassetto:

Nel disegno di legge è riportato che la gran parte delle disposizioni non ha avuto effetto sul rendiconto 2012. Come si è fatto quindi ad arginare il male operato? Massacrando gli italiani di tasse, introducendo in via sperimentale l'IMU, aumentando l'aliquota IVA, le accise e riducendo all'osso le agevolazioni alle imprese. Ma queste vessazioni non sono bastate, perché, malgrado tutto, il debito pubblico è aumentato, come anche gli interessi passivi, che ogni hanno pesano sulle spalle degli italiani e inibiscono ogni margine di manovra per impedire il fallimento del Paese. A questo punto, potremmo essere indotti a pensare che peggio di così non può andare. Leggendo il rendiconto si capisce invece che la situazione è drammatica e che il peggio deve ancora arrivare. Nel 2011, le entrate dello Stato ammontavano a circa 750.000 milioni di euro e le spese a 706.000 milioni;

è successo esattamente l'opposto di quanto avevano preventivato. E attenzione, però, a non farci prendere in giro con il bilancio preventivo, dove entrate e spese vengono volutamente pompate, perché questo consente loro di dire: come siamo stati bravi, abbiamo previsto di spendere di più e invece abbiamo speso meno; avendo speso meno, siamo stati bravi con gli italiani perché li abbiamo massacrati senza pietà di tasse, ma un po' meno di quanto meritavano. Il confronto lo si deve fare con i dati reali, con gli accertamenti e con gli impegni degli anni 2011 e 2012; loro, invece, nelle relazioni pensano di poterci prendere in giro confondendo capre e cavoli. Dal lato della spesa, la situazione è ancora più drammatica: un buco nero che inghiotte tutto. La tendenza è una diminuzione dei contributi di produzione, dell'assistenza alle famiglie e della spesa in conto capitale e un parallelo aumento della spesa per spese correnti e interessi passivi.

Viviamo in un Paese dove 750 miliardi escono dalle casse pubbliche, dove la politica fa passare tra le sue mani la metà del PIL e riesce anche ad indebitarsi, nonostante l'Italia sia uno dei Paesi più tassati al mondo. Nel rendiconto, la missione «Debito pubblico» ha fatto registrare impegni pari al 39,5 per cento del totale della nostra spesa pubblica, di cui solo per interessi passivi si impegna la cifra di 81.000 milioni. Tale voce, nel corso degli anni, è sempre aumentata e le previsioni dei nostri governanti dicono che aumenterà ancora. Ovviamente, le risorse saranno prese riducendo le spese in conto capitale e in ricerca: disprezzano il futuro. Nel frattempo, ci tengono impegnati con le vicende personali di Berlusconi e ci prendono per i fondelli dicendo che aboliranno l'IMU, che come sappiamo verrà sostituita dalla *service tax*; quello che invece nascondono è che per gli italiani il peso del fisco è destinato ad aumentare.

Cito testualmente: «Il peggioramento del saldo netto da finanziare è di 29.187 milioni di euro, quello del risparmio pubblico di 15.512 milioni; il saldo primario peggiora di 29.582 milioni cambiando di segno,

fare solo brevi considerazioni sulle questioni relative, in particolare, al provvedimento di assestamento che è alla nostra attenzione, essendo state analiticamente

sia il rendiconto che l'assestamento mostrano cifre con il segno meno davanti. In particolare, sono diminuite in maniera molto significativa entrate, e i cosiddetti saldi, tutto sommato, sono peggiorati. È chiaro che questo è il segno indotto dalla profonda crisi, non soltanto finanziaria, ma economica del nostro Paese.

89 miliardi, difficilmente rivedibile al ribasso, più probabilmente rivedibile al rialzo. Questo significa che la battaglia per il risanamento dei conti pubblici non deve essere assolutamente in disparte. Il Governo deve sapere che, anche nei provvedimenti in corso, aumenti della spesa pubblica, coperti peraltro con interventi che incidono immediatamente sul mondo produttivo, come le accise, vanno considerati con estrema cautela.

L'aumento secco degli interessi non consente ancora alcun aumento della spesa pubblica che non abbia immediati riflessi nell'attività produttiva. Se, invece, aumentiamo la spesa pubblica corrente e la copriamo con grandezze che incidono sull'attività produttiva non facciamo bene il nostro lavoro. In questo senso, il vero dato positivo che riscontriamo è che comincia a

generale. Le entrate tributarie sono pesantemente diminuite. Questo significa che, al di là di tutte le grida giornalistiche e convegnistiche, le entrate tributarie aumentano solo se aumenta l'attività economica. Tutte le altre questioni si rivelano marginali.

la verità è che il compito su cui dobbiamo insistere è di liberare le attività produttive. Non so quanto dell'area plumbea e grigia che oggi incombe sulle imprese

alla sessione di bilancio, quindi nella sessione di bilancio dobbiamo rivedere bene la questione della liberazione delle forze d'impresa. Penso solo ad una questione, e concludo il Ricordo a tutti i colleghi, della maggioranza e dell'opposizione, che le estreme restrizioni sul contante, che avrebbero dovuto darci non so quali risultati, ne hanno dato uno solo: la riduzione delle attività economiche. Dobbiamo riconsiderare le questioni apertamente. La fotografia è chiara: cresce la diminuzione del PIL (come sapete, era a meno 1,3, poi a meno 1,7, abbiamo accettato meno 1,8, poi vedremo). A ciò è stata correlata immediatamente una riduzione delle entrate tributarie, in particolare sui consumi: ben 10 miliardi in meno di IVA.

offrono una raffigurazione chiara della situazione dei conti e danno chiaro al legislatore l'indirizzo al quale deve uniformare la sua attività, favorevolmente, poco prima della sessione di bilancio ci danno delle indicazioni molto chiare. Sono certo che il Governo proseguirà su questa strada. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore del rendiconto generale

La prima - ed è stata ricordata - anche da altri - è che il rendiconto 2012 offre piena conferma del poderoso e sotto molti aspetti positivo processo di aggiustamento dei conti pubblici realizzato durante lo scorso anno e nella prima parte di quest'anno. Ha comportato ben tre manovre correttive da 81,3 miliardi. Siamo così passati dal possibile *default* finanziario del nostro

soprattutto se si vogliono stilare resoconti di questa fase. È un risanamento certo costoso, che ha determinato l'impennata della nostra pressione fiscale oltre il 44 (era al 42,6 nel 2011), tre punti in più della media europea. Ma l'impennata della pressione fiscale non è stata la sola leva utilizzata, come si continua a sostenere da parte di molti. Se andiamo a vedere i dati del rendiconto, troveremo che un contributo è venuto anche dalla spesa primaria corrente, quella al netto degli interessi: nel biennio 2011-2012 è rimasta sostanzialmente stabile in termini nominali.

Senza sottovalutare la ritrovata credibilità e il ruolo da protagonista recuperato dal nostro Paese in campo europeo e internazionale. Ma è vero che il riposizionamento italiano ha prodotto i maggiori costi per l'economia reale - come sappiamo - con una recessione produttiva e un aumento della disoccupazione così intensi e prolungati come non si era mai verificato - anche in questo A questo ha dato un contributo significativo anche il contesto europeo, prostrato oltremodo da politiche inadeguate perché eccessivamente restrittive.

tra gli otto e i dieci miliardi. Non dimentichiamolo. Il Partito Democratico ritiene che ci sia comunque bisogno di fare altro, di andare oltre la mera austerità e, la sola emergenza dei vincoli. Perché bisogna innanzitutto aggredire le carenze strutturali del nostro Paese che sono alla base del ristagno e delle insopportabili disuguaglianze esistenti nella nostra società.

primo: continuare a ripagare la maggior parte dei debiti della pubblica amministrazione, come si è cominciato a fare. Il secondo: far riaffluire il credito alle imprese,

Allo stesso tempo non si possono continuare ad apporre tagli lineari o semilineari, né si può pensare di aumentare ulteriormente la tassazione. Allora c'è bisogno, per reperire nuove risorse, di una discontinuità profonda nelle politiche pubbliche fin qui attuate. È una strada obbligata e che comporta

che il Governo presenterà in Parlamento entro la metà di ottobre. È in quella sede che andranno presentate le priorità, in anticipo, sia degli obiettivi che si vogliono perseguire sia delle risorse da stanziare per le coperture. Il Partito Democratico si adopererà perché questo appuntamento assuma questa grande rilevanza, proprio per sfruttare l'opportunità della ripresa e favorire l'uscita definitiva dalla recessione.

A questo punto è chiaro che le scelte del Governo nelle prossime settimane saranno decisive per consolidare i segnali positivi, per ora pochi, registrati dalla nostra economia. Potremmo essere realmente a un punto di svolta nella crisi, a patto di non sprecare le opportunità Governo a questo punto e l'instabilità politica che ne seguirebbe produrrebbero costi drammatici, perché rischierebbero di vanificare gran parte dei risultati fin qui raggiunti.

L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro della giustizia sulla riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie». Ha facoltà di parlare il ministro della giustizia, dottoressa Cancellieri. Presidente, signori senatori, come tutti voi sapete tra soli due giorni entrerà in vigore la riforma della geografia giudiziaria. Questa riforma, da tutti ritenuta strategica per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario, è il frutto di un lungo *iter*, iniziato nel lontano luglio del 2011, con il ministro Palma ed il Governo Berlusconi, che vararono la delega, proseguito nel settembre del 2012, con il ministro Severino ed il Governo Monti, che quella delega attuarono con i decreti legislativi nn. 155 e 156. A me ed al Governo di cui faccio parte spetta il compito forse più ingrato: quello di darvi, come la legge impone, effettiva attuazione. Si tratta da lunghissimo tempo attesa, definita epocale durante la cerimonia di inaugurazione dello scorso anno giudiziario dal Presidente della Corte di cassazione, apprezzata dagli studiosi, dall'Associazione nazionale magistrati e dal Consiglio superiore della magistratura; una riforma pienamente condivisa anche da me, dal Governo Letta e straordinariamente sostenuta dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano cui, ancora una volta, va il mio personale ringraziamento. anche di un cambiamento che, facendo venir meno circa il 47 per cento degli uffici giudiziari dell'intero territorio nazionale, suscita, comprensibilmente, vive resistenze nei territori in cui maggiormente incide. Dunque, un intervento costoso in termini di consenso e popolarità, ma che rappresenta un'importante prova di maturità per il Parlamento e per il Governo. Si dimostra così che chi ha il compito di governare è in grado di mettere da parte i propri interessi particolari a favore di quello superiore della funzionalità della cosa pubblica. Se in passato obiettivi come questi sono stati mancati, oggi dobbiamo dimostrare al Paese e a chi ci osserva dall'estero che si è inaugurato un nuovo corso, che guarda al futuro e che tende ad un sistema giudiziario più moderno ed efficiente. Ciò premesso, desidero ricordare che sin dall'esordio del mio nuovo mandato ministeriale ho offerto la piena disponibilità ad ascoltare tutte le sollecitazioni ed i suggerimenti costruttivi finalizzati a migliorare la riforma in Ho, tuttavia, dovuto constatare, non senza rammarico, che l'insieme di tali suggerimenti non si è tradotto in una sintesi unitaria che fosse in grado, senza stravolgimenti, di garantire un intervento integrativo e correttivo largamente condiviso tra le forze politiche. Nel frattempo, la Corte costituzionale rigettando tutti i ricorsi proposti - ad eccezione di quello riguardante il tribunale di Urbino confermava pienamente la validità dei criteri di selezione degli uffici soppressi, sottolineandone sia la ragionevolezza sia la piena conformità alla delega conferita al Governo. Peraltro, le puntuali ed analitiche motivazioni esposte dalla Corte per affrontare le numerose censure sollevate sono, inevitabilmente, destinate a condizionare i limiti, l'ampiezza ed il merito dei possibili interventi correttivi che saremo chiamati a valutare entro i termini previsti dalla stessa legge delega. Basti qui richiamare la riconosciuta ragionevolezza del criterio tramite il quale sono stati soppressi tutti i tribunali con un bacino di utenza inferiore a 100.000 abitanti. Credo che, rimettere in discussione questo criterio - che costituisce uno dei cardini della riforma - significherebbe compromettere l'effettività di quel principio di ragionevolezza riconosciuto dalla Corte costituzionale. Se mi è consentito fare un secondo esempio, anche la proposta di trasformare tutti i tribunali soppressi in presìdi, pur avendo raccolto un buon consenso, non era oggettivamente percorribile, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, l'introduzione di non meglio precisati presìdi di giustizia esula dai limiti di operatività della legge delega. Inoltre, sotto un profilo sostanziale, la surrettizia riproduzione di un modello in tutto sovrapponibile alle sedi distaccate avrebbe, di fatto, compromesso la valenza complessiva della riforma. Tale scelta avrebbe, peraltro, imposto, per ragioni di evidente equità, il riesame, nel merito, della situazione di tutte le altre sezioni distaccate soppresse che, in alcuni casi, vantavano oggettivamente bacini di utenza e carichi di lavoro nettamente superiori perfino alla gran parte dei tribunali soppressi. Detto questo, sono pienamente consapevole che una riforma di queste proporzioni, specialmente in fase di avvio, impone di affrontare non poche difficoltà organizzative, per superare le quali si è fatto ricorso, in numerose casi, allo strumento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 155. Abbiamo ritenuto di utilizzare questo strumento affidandolo, anzitutto, all'iniziativa dei presidenti delle strutture accorpanti. In tal modo, negli ultimi mesi, ho adottato ben 45 decreti ministeriali che, in vario modo e con tempistiche differenti, predispongono le migliori condizioni operative possibili per le situazioni di maggiore criticità riscontrate sul territorio e segnalate direttamente dai capi degli uffici. Ma non ho inteso limitare a questo l'operatività che l'articolo 8 offre al Guardasigilli. Ho ritenuto, infatti, doveroso assumere in prima persona la responsabilità di attivare un'istruttoria finalizzata a valutare, sulla base di criteri rigorosamente oggettivi (bacino di utenza o carichi di lavoro), l'utilizzo degli edifici di alcuni tribunali soppressi, principalmente per lo smaltimento degli affari civili pendenti, per un limitato periodo di tempo. Al termine dell'acquisizione dei prescritti pareri, è mia intenzione adottare un provvedimento *ex* articolo 8 per queste particolari situazioni. Signori senatori, nel concludere il mio intervento avverto il dovere istituzionale di rappresentarvi l'oggettiva impossibilità di fermare, oggi, la riforma. La macchina amministrativa è ormai da tempo avviata: la quasi totalità dei traslochi è già stata eseguita; si sono adeguati i sistemi informatici, trasferita buona parte dei lavoratori interessati, affrontando le spese necessarie. Sono state varate le nuove piante organiche ed il Consiglio superiore - a cui, a partire dal Vice Presidente, onorevole Vietti, desidero rivolgere un pubblico ringraziamento per il sostegno e la collaborazione ricevuti - non ha più coperto i vuoti di organico presso gli uffici soppressi. In pratica, signori senatori, è doveroso che si sappia che tali uffici sono ormai privi di molti magistrati trasferiti ad altra sede, che le nuove udienze sono già pronte per la trattazione nelle sedi accorpanti e che un rinvio - anche di breve durata - produrrebbe con assoluta certezza il caos. Tutto questo, a danno dei cittadini, nell'interesse dei quali la riforma è stata varata. Siamo, dunque, tutti insieme chiamati ad affrontare l'avvio della riforma con spirito costruttivo e lealtà istituzionale, procedendo in corso d'opera al monitoraggio della situazione, per valutare nel prossimo futuro l'eventuale necessità di interventi correttivi entro i termini previsti dalla legge delega. Per questo abbiamo già predisposto, nelle sue linee essenziali, un primo intervento correttivo, con alcune norme organizzative e processuali che renderanno ancor più fluida la fase di avvio della riforma, mentre adotteremo subito dopo anche un secondo decreto correttivo, per apportare alcune modifiche dell'assetto territoriale dei nuovi tribunali, così recependo alcune delle segnalazioni provenienti sia da quest'Aula che dai territori. Sono convinta della necessità di questa riforma e desidero ricordare anche in quest'Aula che il Governo sta operando in linea con le indicazioni formulate dalle istituzioni europee e dalla Banca mondiale che ci invitano a proseguire con decisione in questa direzione. un percorso che, di recente, ha contribuito a far uscire l'Italia dalla procedura di infrazione avviata dall'Unione europea, ma è anche un impegno assunto dal nostro Paese al quale non possiamo e non vogliamo sottrarci.

Signora Ministro, la ringrazio per essere venuta qui in Senato, prima ancora che alcune scadenze diano seguito a questa riforma. Esprimo però - e non non credo solo a titolo personale - molte perplessità sulle comunicazioni che lei ha fatto e sugli atti che sono in corso. So bene che questa vicenda ha attraversato vari Governi ed è stata oggetto di un dibattito che spesso ha diviso al loro interno anche le forze politiche, creando nei nei territori reazioni diversificate a seconda del giudizio o della sorte più fortunata o sfortunata che è capitata a questa o quella realtà. Riteniamo tuttavia che i disagi saranno superiori ai presunti vantaggi di questa riforma. Poiché molti sono i territori in ansia e, anzi, ci sono spesso situazioni di protesta e di disagio che il mondo della giustizia, il mondo forense ed i cittadini stanno esprimendo, non citerò questo o quel caso, almeno personalmente, perché troppi ne dovrei elencare, e le omissioni sarebbero oggetto di risentimento da parte di chi non venisse menzionato. Voglio però ricordare le sue dichiarazioni riferite in particolare ad alcune zone dove i fenomeni criminali hanno una maggiore rilevanza

l'esigenza che, lei stessa, soprattutto per alcune zone d'Italia, aveva giustamente e doverosamente sottolineato. Riteniamo, quindi, che sarebbe giusto tornare su questa materia. Peraltro, il Senato, in data

abbiamo anche votato un ordine del giorno, con un consenso pressoché unanime di quest'Aula, che ci auguravamo potesse servire ad un'ulteriore riflessione e ad un differimento. che decisioni di questa natura impongano poi, in qualche misura, un momento in cui ci si assume una responsabilità; riteniamo però che il servizio della giustizia non sarà avvantaggiato (anche sul piano dei costi è tutto

tutte da dimostrare sul piano dei costi globali, di trasferte e di disagi che i cittadini, il mondo forense e la stessa organizzazione della giustizia in senso stretto dovranno patire e subire. Concludo questo intervento, che non ha voluto citare questo o quel caso perché troppo perché troppo lungo sarebbe stato l'elenco, per manifestare non solo tutte le riserve sui provvedimenti in atto, ma anche l'amarezza per non aver tenuto conto del voto di questa Assemblea, che potrà comunque, con provvedimenti legislativi, dare un indirizzo diverso e alternativo rispetto a quello che, in modo incauto, sta perseguendo perseguendo questo Governo.

non è un corpo estraneo a questo Parlamento: lei è qui e deve riferire al Parlamento, ma deve anche accogliere i suggerimenti che da esso le vengono, e sa perfettamente che la questione relativa alla riorganizzazione degli uffici giudiziari non rappresenta una novità per le Aule parlamentari. Si tratta infatti di un tema che tiene banco da diversi mesi, e che ha visto avvicendarsi al Dicastero della giustizia ben tre Ministri. Questo, solo per parlare dei tempi più recenti, perché a ben vedere è da circa un decennio che si parla della necessità di razionalizzare gli uffici giudiziari, senza che fino ad oggi si sia riusciti a portare a casa alcun risultato apprezzabile. Ritengo infatti che i bacini di utenza, il carico di lavoro e lo stato degli edifici siano importanti,

credo ormai sia in coma profondo, sia da rianimazione e necessiti di una considerazione un po' più attenta. Alla luce di queste considerazioni, tenuto conto che la questione incombe sul tavolo politico con una certa pressione da almeno due legislature, ritengo sia importante fare tesoro non solamente degli sviluppi

allorché fu sottoposto al parere del Parlamento lo schema di decreto legislativo recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero». Proprio sullo schema in questione vi fu infatti una soddisfacente quanto sofferta convergenza politica in Commissione giustizia del Senato, che non sarebbe giusto ignorare. D'altronde, la sovranità popolare, signor Ministro, è qui, e se la Commissione converge su punti ben precisi, perché il Ministro non li tiene in considerazione? Perché il suo predecessore non li ha tenuti in considerazione? Quali interessi aveva? Quali *lobby* doveva difendere il suo predecessore? prima della pausa estiva, come riferiva poc'anzi il senatore Gasparri, quest'Aula ha approvato un ordine del giorno con cui si impegnava il Governo a tenere conto proprio delle direttrici emerse nel corso della passata legislatura in entrambi i rami del Parlamento, frutto di un fitto lavoro e di una sintesi politica di cui oggi sarebbe quanto meno inopportuno non tener conto. Lei, signora Ministro, non può non tener conto della volontà di quest'Aula, altrimenti è una perdita di tempo. Cosa votiamo a fare gli ordini del giorno che il Governo accoglie e poi non tiene in considerazione? Non sarà per caso caso in scacco di *lobby* che all'interno del suo Dicastero le impediscono di portare avanti la volontà di questa Assemblea? Lei non può non tener conto di quanto questa Assembla ha votato. Anche nel corso dell'attuale legislatura la questione della cosiddetta geografia giudiziaria giudiziaria è sbarcata tra i banchi della Commissione giustizia, di cui faccio parte, che pressoché all'unanimità ha votato una proroga dell'entrata in vigore, che dovrebbe avvenire dopodomani, del provvedimento che prevede la soppressione di 30 tribunali, 30 procure, 220 sezioni distaccate e 667 sedi di giudici

in Commissione giustizia è un rinvio teso non ad accantonare il provvedimento bensì ad addivenire ad un testo che abbia come immediata conseguenza un efficientamento dei tribunali, oltre che la razionalizzazione degli uffici giudiziari. L'efficienza della giustizia, signor Ministro, è sinonimo di civiltà è deve essere, quindi, l'obiettivo cui mirare. Questo è il risultato che noi tutti dovremmo voler portare a casa, partendo da alcuni capisaldi, come ad esempio la durata dei processi che - lo dico apertamente - non può essere barattata per principi basati meramente sull'economicità. Dico questo perché, se volessimo basarci esclusivamente su un principio che imponga un'ottica tesa al risparmio, il primo passo da compiere non dovrebbe essere quello di intervenire sul settore della giustizia ma sulla mala giustizia, che rappresenta un costo enorme per lo Stato pari a circa un punto e mezzo di PIL l'anno (e sto parlando di 20-25 miliardi l'anno). Se dunque la fretta di approvare celermente un provvedimento volto a chiudere un certo numero di tribunali è dovuta alla necessità di fare cassa, mi dispiace ma siamo fuori strada, perché è sul funzionamento o, meglio, sul cattivo funzionamento di tutta la macchina della giustizia che bisognerebbe intervenire. La giustizia in Italia è malata e deve essere I magistrati che occupano posizioni di potere nei vari Ministeri, e in quello della giustizia in particolar modo, dovrebbero essere sostituiti, forse da medici o sciamani che curino questa malattia che affligge il Paese. A tal proposito, le ricordo come attualmente, nonostante un *referendum* del 1987 puntualmente ignorato, la riparazione dell'errore giudiziario sia a carico dello Stato perché, contrariamente a quanto manifestamente espresso dagli italiani nella richiamata consultazione referendaria, ci si continua a rifiutare di introdurre nel nostro ordinamento la responsabilità civile dei magistrati, cosìcché, mentre qui si discute di come risparmiare quattrini ridimensionando il numero dei tribunali - cosa giusta, per carità - lo Stato e per esso i cittadini continuano a sovvenzionare gli errori giudiziari e, per di più dal momento in cui questo provvedimento entrerà in vigore, avranno maggiori difficoltà e dovranno affrontare costi maggiori per raggiungere le sedi giudiziarie che resteranno in essere. In un'ottica di razionalizzazione della spesa corrente, estendere anche alla magistratura il principio valido per qualsiasi altra categoria di professionisti che sono obbligati in solido dinanzi all'errore da essi compiuto, non sarebbe un primo passo? Immaginare di far procedere parallelamente la razionalizzazione delle sedi giudiziarie e la soluzione all'annoso problema del sovraffollamento carcerario - che ci costa sia in termini di risarcimento danni che di potenziali non sarebbe più logico in un discorso organico di efficientamento di un servizio nell'ottica dell'economicità? L'Unione europea ci ha dato tempo fino a maggio 2014, signora Ministro: ricorderà questa data. La razionalizzazione delle sedi giudiziarie è importante, ma è prioritaria rispetto alla condizione in cui versano persone che in pochi metri quadrati trascorrono la quasi totalità delle proprie giornate, stando letteralmente l'una addosso all'altra, spesso con scarsa luce ed aria? Mentre la Corte europea dei diritti dell'uomo richiama l'Italia affinché venga ripristinata la legalità all'interno dei penitenziari,

al seguito delle proprie madri detenute, secondo i dati al 31 agosto, rappresentano un costo? In un'ottica di razionalizzazione della spesa, obiettivo del provvedimento in discussione, cosa si pensa di fare in tal senso? Sia chiaro, questo provvedimento deve vedere la luce al più presto, ma non si possono ignorare le istanze sollevate nelle Aule parlamentari, nelle Commissioni di merito, ma soprattutto dai cittadini, per i quali la giustizia non può rappresentare un costo ulteriormente maggiore rispetto a quello attuale il termine «costo» non intendo richiamare solamente aspetti economici). Per questi motivi il provvedimento non dovrà discostarsi dalla delega ricevuta nella scorsa legislatura, i cui parametri nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere erano tali da considerare, tra gli altri, la la «specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale» ed il «tasso di impatto della criminalità organizzata». In ballo ci sono dunque costi, sia in termini economici che sociali, i quali imporrebbero un'accurata riflessione sull'opportunità di mantenere in essere, nelle sedi dei tribunali soppressi, una sezione distaccata del tribunale accorpante, così da assicurare un'adeguata e funzionale presenza di uffici giudiziari sul territorio, per garantire gli indispensabili fini di efficienza della macchina giudiziaria. In conclusione, signora Ministro, la riforma della geografia giudiziaria nei termini in cui è stata posta in essere andrebbe collocata,

che noi abbiamo del precedente ministro Severino credo sia tale che la invitiamo a rivedere e

una piccola premessa. Noi componenti del Gruppo Autonomie e Partito socialista italiano siamo del parere che questa riforma debba andare avanti. avanti. È una riforma per certi versi coraggiosa; non deve essere però l'unica che riguarda la giustizia, ma deve essere una riforma che raggiunge gli obiettivi che ha dichiarato: gli obiettivi che ha dichiarato: rispondere all'esigenza di contenimento dei costi, aumentare l'efficienza e quindi portare ad una svolta nel nostro Paese per quanto riguarda questa annosa questione.

depotenziarla negli effetti pratici e nella percezione dell'opinione pubblica, che la vede soltanto come ulteriore penalizzazione dei propri diritti, del proprio diritto ad avere un servizio di giustizia adeguato, efficiente, rapido e vicino alle proprie realtà territoriali. Perché vicino alle proprie realtà territoriali? Signora Ministro, non si tratta di esercitare un'azione di ammodernamento e razionalizzazione del nostro sistema se i costi vengono spostati dal bilancio dello Stato al bilancio delle famiglie.

che avvicina i cittadini a questo Stato, molto spesso distratto sugli interessi generali e molto attento alle situazioni particolari. Per carità di Patria non tocco l'argomento all'ordine del giorno in altra sede,

Un esempio è la soppressione dei tribunali di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi. un territorio che, con l'attuazione della riforma, dal 13 sarà privato della presenza dello Stato in un servizio essenziale per una zona incrocio di organizzazioni criminali mafiose interregionali, 'ndrangheta, sacra corona unita, camorra e quant'altro la fantasia criminale del nostro Paese ci mette a disposizione. Non possiamo privare quel territorio di un servizio. È un territorio quasi equivalente a quello di una Regione contigua, la Basilicata.

Non è pensabile accorpare Rossano su un tribunale certamente minore, che ha la sua dignità di tribunale ma che è molto distante rispetto a quella realtà. Per Lucera vale lo stesso ragionamento di Rossano Ma voglio portarmi in altre aree, signora Ministro. Voglio riferirmi ad aree più vicine alla mia realtà territoriale. Mi riferisco alle problematiche della Liguria. Ci sono tribunali che hanno grandissime problematiche criminali e che vengono soppressi e altri la cui competenza

ma di esercitare una semplice azione con un pennarello di colore rosso: spostare un confine geografico di giurisdizione tra un territorio ed un altro. È l'esempio della mia realtà. Parlo di questo perché

dove passa un treno ogni ora e mezza, quando orino è servita da decine e decine di autobus, metropolitane e quant'altro. Signora Ministro, spostare la competenza dell'ex sezione distaccata di Chivasso su Ivrea, se non quella di favorire operazioni corporative? È inaccettabile, questa non è riforma della giustizia. Signora Ministro, non voglio utilizzare tutto il tempo a mia disposizione. Il peso della responsabilità che sento sulle mie spalle mi induce ad aumentare il tono della voce, ma non voglio assolutamente farlo perché lei merita tutto il nostro rispetto e la nostra attenzione; noi confidiamo nella sua sensibilità e volontà di rimuovere questi problemi. Ci aspettiamo che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, come ha detto lei, si possano attuare le modifiche dell'impostazione attuale per dare attuazione al principio del rispetto della volontà popolare, che oggi qui rappresentiamo. Oggi, signora Ministro, le diciamo con il cuore in mano che c'è bisogno di fare la riforma,

Onorevole Ministro della giustizia, vorrei richiamare la sua attenzione sulla mancata inclusione della sezione distaccata di Ostia tra le sedi giudiziarie che rimarranno aperte per due anni per lo smaltimento dell'arretrato. Per tale sede giudiziaria ricorrono infatti tutti i presupposti da lei stessa posti alla base del recente decreto con il quale è stata autorizzata la continuazione dell'attività, per un periodo di due anni, per ben otto tribunali. Si ritiene che sia un grave ed imperdonabile errore non autorizzare la continuazione dell'attività anche all'ufficio giudiziario di Ostia, del quale occorre tenere presente la specificità del contesto territoriale ed il bacino di utenza. Infatti, la sezione distaccata di Ostia ha competenza sul territorio del X municipio di Roma Capitale (ex XIII), di circa 300.000 abitanti effettivi,

come parametro di riferimento per la selezione dei tribunali da lasciare aperti per lo smaltimento delle pendenze. Né può valere come giustificazione per la mancata inclusione di Ostia la circostanza che trattasi di sezione distaccata, perché il Ministro conosce bene che l'area metropolitana di Roma - che da sola presenta una popolazione maggiore dell'intero circondano di Milano - ha posto più volte l'esigenza di istituire un secondo tribunale all'interno del Comune capoluogo, come del resto è accaduto per Napoli, e di ciò già si discusse nella relazione al primo decreto legislativo n. 491 del 1999 di revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Pertanto, la peculiarità della sezione distaccata di Ostia, permettendo il decongestionamento dell'ufficio giudiziario di Roma che presenta le maggiori dimensioni a livello europeo, giustificherebbe una soluzione diversa da quella adottata per le altre circoscrizioni e sedi distaccate di tribunale. Al fine del rilevamento, inoltre, del secondo valore soglia da lei posto per la continuazione dell'attività per ulteriori due anni, cioè quello relativo alle sopravvenienze, è risultato da un'indagine comparativa che la sezione distaccata di Ostia ha carichi di lavoro maggiori di quelli di veri e propri tribunali dei quali lei ha recentemente decretato la permanenza. Ciò costituisce un'ulteriore prova della necessaria differente soluzione da adottare per Ostia rispetto alle altre sezioni distaccate e costituisce prova di un'inaccettabile ed inspiegabile disparità di trattamento tra l'ufficio giudiziario di Ostia e gli otto tribunali lasciati aperti. L'ufficio giudiziario di Ostia ha dimostrato, inoltre, un'esemplare efficienza, con indici di smaltimento altissimi, che hanno prodotto nel biennio 2010-2011 caso unico nel distretto di Roma, anche per l'utilizzo intenso della mediazione delegata - un decremento delle pendenze del 32 per cento, come attestato dal presidente della corte d'appello di Roma nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2012. Ma ciò che più di tutto mi preme sottolineare, onorevole Ministro, è che questo tribunale opera attivamente in un territorio ad alto rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata - come le cronache attestano da tempo - con porto, aeroporto e traffico di stupefacenti, condizione che rende particolarmente importante la presenza *in loco* di un presidio dello Stato, dove si celebrano convalide di arresti e processi penali anche nei confronti della manovalanza della criminalità organizzata. Chiudere il presidio di giustizia sul litorale romano comporta un reale arretramento dello Stato con abbandono del territorio. Va infine sottolineato che nella legge delega il principio direttivo di primaria importanza nella revisione della geografia giudiziaria è quello della razionalizzazione del servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane, tra cui Roma, che deve essere necessariamente realizzato mediante decongestionamento del tribunale metropolitano. Quindi l'obiettivo della riforma appare palesemente stravolto dalla soppressione delle sezione distaccata di Ostia che imporrebbe di riversare sull'unico tribunale metropolitano il carico di lavoro dell'ufficio soppresso, con ciò determinando un ulteriore congestionamento di uffici già oltremodo gravati. In conclusione, si ritiene che ci siano tutti i presupposti, vista la specificità dell'ufficio giudiziario di Ostia al confronto con le altre sezioni distaccate, per concedere una proroga di due anni, con la consapevolezza che tale soluzione avrebbe comunque carattere parziale rispetto ai gravi problemi che affliggono la giustizia della Capitale, ma che può servire a porre mano ad una diversa soluzione normativa che istituisca un secondo tribunale cittadino, come è avvenuto per Napoli. La invito pertanto, onorevole ministro Cancellieri, a considerare tale opportunità e ad includere l'ufficio giudiziario di Ostia tra i presidi di giustizia da lasciare aperti per ulteriori due anni al fine di smaltire i procedimenti pendenti.

È quanto ci è stato segnalato dagli ordini degli avvocati, dai tribunali e dai Comuni: non si tratta di un miglioramento dell'efficienza. Ci sono dei problemi gravissimi che sono stati evidenziati.

della proroga: ogni volta c'è sempre stato un procrastinarsi della situazione, sempre nell'attesa che venissero questi decreti correttivi. Se era così convinta che non si dovessero adottare decreti correttivi, dal momento che la riforma doveva essere fatta così,

Il sospetto viene anche perché, sempre nell'ambito di questo arcano procedimento, in Commissione giustizia abbiamo deliberato sulla proroga e l'abbiamo approvata a maggioranza, mentre, poi, i primi di agosto,

Potevamo benissimo approvare qui la proroga, se è vero che il Parlamento lo voleva, come si continua a sentir dire sui *media*. Sento anche i rimproveri mossi dalla maggioranza nei confronti del Governo.

Se è vero che il Parlamento voleva una cosa, che è stata espressa nei pareri al Senato e con gli ordini del giorno (non solo quello della Lega, che è stato accolto, ma anche quello del PD, che è stato votato

questi decreti correttivi. Ormai la frittata è fatta, i problemi sono già in corso. Chi lavora dentro i tribunali si rende conto di cosa vuol dire. Adesso è entrata in vigore la riforma: come si fa a tornare indietro? Come si fa, dopo che si è fatto un trasferimento o una soppressione, a tornare indietro? C'era il tempo. Da quando è cominciata questa legislatura ad ora c'era il tempo, quindi è inutile che la maggioranza continui ad alimentare le speranze. La frittata è fatta, gli errori sono stati commessi, è entrata in vigore questa riforma e i problemi si sono creati. Spero che poi, con gli anni, ci si accorga che magari qualcosa potrà anche aver portato buoni frutti.

con il quale, per alcuni tribunali, viene concessa una forma di proroga per poter esaurire delle cause pendenti, limitatamente ad alcuni settori? Ciò crea un ulteriore pasticcio. Questo lo vedono: qui in Aula ci sono delle persone che ci stanno lavorando. Sono qui in tribuna e ci stanno guardando; sanno cosa vuol dire lavorare in un tribunale, i problemi che crea anche questo decreto ministeriale.

signora Ministro, dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi e in previsione di quelli che ascolterò, conoscendo dei prossimi oratori la personalità, l'appartenenza e le opinioni che hanno espresso in questa sede e altrove, ci troveremo quasi soli con le nostre buone ragioni a essere completamente d'accordo come Gruppo e come persona con la sua iniziativa e con la coraggiosa decisione che ha adottato. Come spesso accade a tutti noi quando ci troviamo di fronte a dei contrasti, quando dobbiamo vivere il conflitto di opinioni diverse, la difficoltà di decidere in quello che crediamo giusto e magari anche opportuno, ci accade di rievocare qualcosa di nostro, di intimo, le convinzioni che hanno fatto la nostra educazione, i valori in cui crediamo. Mentre ascoltavo parlare lei, con le difficoltà che ha incontrato nel sostenere questo provvedimento e le contrarietà in questa sede, nei territori e nel dialogo con le varie corporazioni di appartenenza si sono frapposte a questa decisione, mi sono venute in mente due citazione latine; mi consentirete la civetteria di rievocarle. Una è il motto di un mio amico e maestro, un gesuita, cardinale di Milano: *pro veritate adversa diligere*. Un altro è un motto che mi hanno insegnato i padri gesuiti (scuola che ho frequentato per dodici anni) e che viene applicato di solito per sostenere i contraddittori, ma che in questo caso vale anche per le decisioni politiche (e mi sembra che lei, pur non avendo frequentato la scuola dei gesuiti, non potendolo fare come

Lei lo ha applicato integralmente, rigida nei principi di applicazione e duttile nei comportamenti per adottarlo. impedire agli altri di criticarlo, farò una breve esposizione del perché consideriamo questo provvedimento necessario, ancorché contrastato e di difficile applicazione, pur suscettibile degli aggiornamenti e dei miglioramenti che il percorso funzionale consentirà. Forse non tutti sanno che il Forum economico mondiale ha definito il nostro Paese, nella graduatoria dell'efficienza del sistema legale nel definire le controversie, al 145° posto sui 148 che sono stati considerati. I parametri di riferimento per l'efficienza nel definire le controversie concernono la durata dei procedimenti e la prevedibilità, in base al diritto scritto, alla legge vigente, delle decisioni. è stato ampiamente affrontato anche dall'OCSE e dal Fondo monetario internazionale il criterio del sistema giudiziario efficiente come uno dei fattori principali per la competitività di un Paese. Il nostro sistema giustizia è minato alla radice da una durata eccessiva, da una farraginosità delle procedure, da una articolazione - e veniamo al punto che ci riguarda della geografia giudiziaria, che data intorno, se non vado errato, alla seconda metà dell'Ottocento. Potete immaginare le condizioni che si sono modificate da allora ad oggi le diseconomie organizzative e i costi eccessivi che questo sistema fisso, in un quadro cangiante, in una complessità sociale ed economica così in evoluzione, ha determinato. In effetti, gli studi fatti sull'efficienza dei tribunali hanno dimostrato che, come accade nell'economia italiana, sono le medie imprese, più ancora delle piccole o delle grandissime, che sanno essere efficienti. È stato infatti dimostrato che gli uffici giudiziari che funzionano meglio sono quelli che hanno un organico che va dai 30 ai 60 magistrati, con relativi interventi a supporto della struttura di personale amministrativo. È questo il criterio che ha ispirato l'intervento perché se da un lato sono stati chiusi i piccoli uffici giudiziari, quasi inconsistenti nelle loro dimensioni, che però avevano un costo strutturale e organizzativo elevato,

La Corte costituzionale - lei, signora Ministro, l'ha citata - aveva dato delle indicazioni per l'applicazione di questa norma, che lei ha puntualmente rispettato nel prendere questa coraggiosa decisione. Vorrei fermarmi anche su un altro punto, che è una conseguenza ortogonale della diversa distribuzione, della razionalizzazione di questi interventi, non prevede solo la chiusura di alcuni tribunali e l'accorpamento di altri, in base a parametri molto lucidi e oggettivi, ma anche, in conseguenza di questo, una diversa distribuzione delle piante organiche. Infatti, nel momento in cui le sedi vengono ridisegnate in termini più razionali

professionalità giurisdizionali, cioè dei magistrati, sia del personale amministrativo, così come la specializzazione di alcuni tribunali per competenze specifiche, possono essere meglio organizzate. È con queste considerazioni-quadro che, pur in presenza delle criticità che tutti riconosciamo, vogliamo dare il nostro contributo convinto, determinato e assolutamente coerente alle decisioni che lei, signora Ministro, e il Governo in carica, a cui diamo il nostro sostegno, avete adottato, consapevoli

si potranno affrontare le criticità e rimodularle. In proposito, lei ha infatti citato nel suo intervento introduttivo già due provvedimenti in allestimento per perfezionare l'insieme su dati esperienziali. A quel punto vedremo, come accade spesso in molte altre circostanze, che le criticità che sono state palesate, a volte con un pregiudizio, saranno superate dal giudizio di efficienza, non solo economica, ma anche funzionale, che un buon funzionamento degli uffici giudiziari consentirà

Grazie, signora Ministro, per il coraggio che ha dimostrato. Lei ha la nostra adesione. Non saremo numerosissimi, ma i fatti sono testardi.

nel ricordare le numerose criticità, perplessità e valutazioni assolutamente negative riferite a come questo piano di riordino della geografia giudiziaria avrà ingresso nelle nostre aule da qui a due giorni.

noto. Infatti, come sappiamo, in Commissione giustizia sono mesi che vi è una interlocuzione, soprattutto da parte di esponenti delle forze della maggioranza che sostengono il suo Governo, in merito all'opportunità

di riordino e cosa starà accadendo in tutta Italia, dal Nord al Sud. Forse sono troppo pessimista, non lo so, staremo a vedere. Anche a me piacerebbe unirmi all'afflato ottimistico del senatore Albertini, così come al richiamo della senatrice della Lega, Lega, che spera che in corso d'opera si possa aggiustare e migliorare il testo. La verità è che il mio, il nostro pessimismo sembra essere fondato sulla scorta di considerazioni che lei probabilmente non ricorderà, perché chissà quante voci avrà ascoltato, molto più autorevoli della mia, della nostra. Non so se ricorda un'audizione svolta il 28 maggio scorso in Commissione giustizia del Senato,

allora riferimento a una circostanza che è poco nota e che mi piace ricordare, per i presenti e per chi ascolterà queste parole in seguito:

Il Governo Monti, sostenuto - ricordiamolo - dalle medesime forze che oggi compongono l'attuale Governo, in relazione ai costi della giustizia civile e amministrativa indicava che: «Al fine di decongestionare i tribunali, il Governo ha aumentato la tassazione sia sui procedimenti di secondo grado e di Cassazione sia sul processo amministrativo. Da gennaio 2013 è raddoppiato il contributo unificato per le impugnazioni che sono respinte. È introdotto un controllo preliminare di ammissibilità sulla richiesta d'appello. Se l'impugnazione è dichiarata inammissibile o improcedibile, è prevista una sanzione a carico della parte proponente. In tal caso, il compenso dovuto al legale è ridotto della metà».

la nuova geografia giudiziaria è l'ulteriore tassello che darà forse il colpo di grazia al sistema giustizia già morente - ovvero sostanzialmente la desertificazione della giustizia, frapponendo ostacoli fra il cittadino e la richiesta di tutela dei propri diritti, tutela garantita nominalmente dall'articolo 24 della Costituzione, quali l'aumento dei costi (il contributo unificato è la tassa che si paga per intentare azioni civili), la delega ad organismi privati della mediazione obbligatoria e trappole procedurali che poco hanno a che fare con l'ottenimento di una sentenza intrinsecamente più giusta, mere trappole procedurali con cui avvocati e magistrati dovranno

del Governo e del Parlamento senza pregiudizi di tipo ideologico, approvando quello che condividiamo e opponendoci con il massimo delle nostre forze in caso contrario. Questo è uno dei casi in cui

i partiti della maggioranza non sono riusciti ad imporre la voce della ragionevolezza nei confronti del Governo che loro sostengono. Come è possibile? Cosa sta succedendo? In quale Paese viviamo?

quanto meno in tema di giustizia, è volta alla risoluzione dei problemi semplicemente desertificando la giustizia e rendendo più difficile difendere i propri diritti in sede civile e scaricando sui privati i maggiori costi

*(PdL)*. Signora Ministro, credo dobbiamo ricordare a tutti che la Repubblica italiana è una Repubblica parlamentare che vede al centro delle istituzioni il Parlamento.

nel senso che io credo fortemente nella necessità di un dialogo costante tra Parlamento e Governo, purché non sia formale, ma sia sostanziale, che abbia la capacità di individuare strumenti, modalità di interventi che abbiano la capacità di convincere.

le ragioni alla base della modifica delle circoscrizioni giudiziarie voluta dal Governo Berlusconi e, in particolare, dall'ex ministro Palma.

tra Governo e Parlamento. Infatti, volevo evitare interessi campanilistici; volevo evitare la discrezionalità e garantire efficienza al sistema complessivo. dal senatore Albertini fanno vergogna al nostro Paese. Allora, bisognava creare un sistema di efficienza e di minori costi. Il sistema creato determinerà maggiori costi e minore efficienza. Con lo stesso spirito, smessi i panni di rappresentante del Governo, sono venuto in Parlamento e ho lavorato in Commissione giustizia con gli altri senatori

fatto riferimento ai criteri per ottenere maggiore efficienza. Signora Ministro, negli anni Settanta in Francia furono effettuati studi di docimologia per verificare quali erano i tribunali con maggiore efficienza. Un ufficio giudiziario

e per circa diciotto sezioni distaccate. Lei sa meglio di me che il provvedimento della Commissione giustizia riguardava quegli otto tribunali e in tutto trenta sezioni distaccate. (è bene che si sappia), lei aveva l'accordo totale, unanime del Parlamento per l'eliminazione degli uffici dei giudici di pace su 190 sezioni distaccate, su 19 tribunali.

come arrivare alla soluzione di individuare una competenza diversa che fosse di maggiore efficienza. Oltre agli otto tribunali, c'era ancora Crema

Rispetto a queste situazioni non si può pensare di scaricare i costi e dire che risparmieremo. Signora Ministro, ho molta fiducia in lei, perché la conosco da quando era alla prefettura di Milano.

faccio due esempi: quanto costa la riconversione del tribunale di Chiavari, e quanto costa la riconversione del tribunale di Bassano del Grappa? Ce ne sono però anche altri. Non voglio dire ciò che costerà in termini di traduzione abolire

Nessuno le ha chiesto di salvare il tribunale di Chiavari così com'è; le abbiamo chiesto di salvare il tribunale di Chiavari, ma di spostare la competenza fino a Genova, perché ciò significava diminuire il lavoro di Genova e avere due funzionari forti ed efficienti. Nello stesso tempo, avremmo avuto un tribunale di ultima costruzione attaccato al carcere. Sono cose che non le devo dire. Non abbiamo avuto risposta. Perché? La grandezza degli uomini si misura nel momento in cui si torna indietro e si ha la capacità di ammettere che c'è la possibilità della correzione. *(Applausi dal Gruppo PdL e

è conosciuto perché ha un'enorme difficoltà a fare le riforme, e questo ci viene rimproverato anche dagli organismi internazionali, anche nel settore della giustizia. Il nostro Paese ormai non può più fare a meno delle riforme: il Paese uscirà fuori da questa crisi se la userà come un'opportunità storica, senza precedenti, per realizzare quelle riforme attese da anni. E quella delle circoscrizioni giudiziarie era una riforma attesa da due secoli.

l'applicazione delle riforme. Anche in questo il nostro Paese ha un limite strutturale. Il nostro Paese, anche quando vara delle buone riforme, al momento della loro applicazione si perde.

e le proposte che le avanziamo si pongono alla luce di questo secondo aspetto: vogliamo che questa riforma sia applicata bene e che sfugga a quella maledizione dell'Italietta

una misura moderna e avanzata nella riorganizzazione degli uffici giudiziari. Ministro, erano cinque i criteri da seguire per una buona lei li conosce bene: numero degli abitanti, carichi di lavoro, indice delle sopravvenienze, (attenzione, Ministro) specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, infrastrutturale, e un quinto criterio, per me forse il più importante, presenza di criminalità organizzata. Ministro, mancano all'appuntamento con l'applicazione della riforma questi due criteri, quello su cui chiedevo una sua particolare attenzione. Guardi con onestà intellettuale, Ministro (che lei ha, che le è riconosciuta), ai cinque criteri e scoprirà che gli ultimi due non sono stati tenuti in considerazione in modo serio né nel decreto attuativo né, adesso, nelle misure che lei ha ritenuto di favorire con l'articolo 8

Un numero limitato, con motivazioni oggettive, in coerenza con i parametri previsti dalla legge delega sulla riforma. Questo ancora non è avvenuto, e noi continuiamo ad avanzare quella

tant'è vero che in qualche caso con l'articolo 8 si è dovuto limitare l'applicazione della riforma. Allora, piuttosto che aspettare un risultato negativo, un moderno Paese prevede, analizza, progetta, organizza e fa in modo che tale

poteva utilizzarsi la soluzione di trasformarli in sezioni distaccate. Signora Ministro, guardi che la proposta dei presidi non è mai nata dal Parlamento: è un'idea balzana, lo condivido, forse anche un po' ridicola, nata negli uffici del Ministero della giustizia. Non era neanche una sua proposta. Ecco perché l'argomento, che lei giustamente ha criticato, dei presidi giudiziari non era da rimproverare al Parlamento: è un argomento che lei deve utilizzare per rimproverare i suoi uffici. Noi le abbiamo chiesto, anche qui con parametri certi e oggettivi, di tenere in piedi poche sezioni distaccate, in condizione di offrire al territorio un moderno servizio della giustizia: avanzato, consapevole, intelligente, efficiente. efficiente. Devo ringraziare i parlamentari del mio Gruppo, 108 senatori, perché non hanno avanzato nessuna richiesta localistica. Sono stati capaci di esercitare il loro mandato parlamentare, di interloquire con il territorio, ma di non farsi prendere dalla logica della vandea localistica. Ed hanno avanzato soluzioni che l'hanno raggiunta direttamente e con atti formali per correggere l'avvio di questa riforma e rimetterla in coerenza con i parametri previsti dalla legge delega.

Quando siamo scesi nel concreto la stessa Scelta Civica ha condiviso molte delle nostre soluzioni. Ministro, non abbia paura del Parlamento: è una risorsa è una risorsa democratica e nel merito di questa riforma ha avanzato proposte serie. Prima della chiusura dei lavori per la pausa estiva, proprio un mese fa, ha approvato un ordine del giorno sottoscritto da tutti i che avanzava proposte molto serie; per cui, si fidi di questo Parlamento, lo ascolti, perché qui non c'è nessuna voglia di stravolgere la riforma. C'è la necessità di ascoltare il territorio, di adottare le soluzioni più avanzate e più coerenti e di interloquire con il Governo per fare in modo che l'Italia, per la prima volta, sappia non solo varare la riforma, ma anche applicarla bene e con coerenza. Signora Ministro, i decreti correttivi sono nella sua disponibilità, sono previsti dalla legge. Il Parlamento, naturalmente, adesso dovrà decidere come portare avanti le proprie istanze. Noi faremo di tutto per evitare che vengano iniziative di legge sui singoli tribunali perché si mantenga un progetto di coerenza, ma lei faccia in modo che con i decreti correttivi si eviti questa deriva

Ringrazio il ministro Cancellieri per la sua disponibilità. Sono certo che sarà sensibile a tutte le sollecitazioni venute dall'Assemblea e da tutti i Gruppi parlamentari.

Tuttavia credo che la maggioranza di noi non sia coerente: anzi, non siamo neanche seri. Questo Paese non cambierà mai se andiamo avanti così. Noi non siamo coerenti, perché ci sbracciamo tutti nei comizi, nelle piazze e nei dibattiti televisivi a parlare di modernizzazione, di riduzione dei costi, di cambiamento dell'Italia, di rinnovamento. Poi, quando siamo alla prova dei fatti ci comportiamo in maniera diametralmente opposta. Non siamo coerenti. Non siamo seri. Non vogliamo modernizzare il Paese. Quando siamo alle prese con una questione vera, facciamo un passo indietro.

È un problema che riguarda anche noi, sulla nostra pelle, riguarda il nostro Presidente, il nostro Gruppo parlamentare, il nostro partito. Pensiamo davvero che il problema della giustizia in Italia sia costituito dalle sedi distaccate?

Per quanto mi riguarda, a titolo davvero personale, le dico, signora Ministro: lei è una persona seria, vada avanti. Faccia qualcosa di buono e di serio per tutti gli italiani e per questo Paese, che ne ha davvero bisogno. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle richieste di adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento per il disegno di legge n. 119, concernente su tali richieste l'Assemblea delibera senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse soltanto le dichiarazioni di voto.

la posizione della Lega Nord sui parchi è molto diversa da quella del disegno di legge n.119, di cui oggi siamo chiamati a votare la dichiarazione d'urgenza, teso a modificare la legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991. Tengo a premettere e sottolineare che la Lega Nord è a favore di tutte quelle azioni che contrastano la tendenza alla perdita della biodiversità, attraverso la tutela delle aree protette e degli ecosistemi. Questo sia per ottemperare agli obiettivi fissati in sede comunitaria e internazionale, sia per la stessa conservazione della specie umana, sulla cui salute studi scientifici dimostrano come incida positivamente la stabilità degli ecosistemi. Il nostro Paese detiene il primato europeo nella biodiversità, ha una dotazione importante di *habitat*, molti di questi dichiarati prioritari a livello comunitario. Tra parchi nazionali e regionali e aree marine protette, risulta tutelato circa il 12,5 per cento dell'intero territorio nazionale: una percentuale che, se sommata ai SIC (siti di interesse comunitario) e alle zone di protezione speciale, arriva quasi al 22 per cento. Si tratta di una risorsa che occorre adeguatamente valorizzare e non trattare come un mero vincolo territoriale.

da anni, bensì un'opportunità di sviluppo, anche ai fini turistici, e di preservazione delle tradizioni e delle identità dei territori. La Lega Nord ritiene, come abbiamo ribadito in sede di trattazione delle mozioni sul dissesto idrogeologico, che le Regioni e gli enti locali devono assumere un ruolo chiave non solo per la tutela delle acque, per la difesa del suolo e delle zone a rischio, ma anche per la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Per noi le Regioni e gli enti locali, ossia le istituzioni più vicine alle necessità del territorio e alle comunità dei cittadini, devono essere i soggetti responsabili della *governance* delle aree protette e della co-pianificazione paesaggistica, secondo strumenti di regolazione non limitati a vincoli e divieti, ma rivolti verso forme attive di utilizzazione del territorio e di coinvolgimento della popolazione. Per noi il permanere delle aree protette nazionali risponde oramai ad esigenze di mero finanziamento delle spese correnti degli enti parco e, vista l'esiguità delle risorse disponibili, interessa solo quegli enti meno virtuosi che non sono in grado di sviluppare finanziamenti mediante idonee pratiche di autofinanziamento, di sviluppo del turismo sostenibile e di promozione dei prodotti tipici. Siamo convinti che occorra un radicale ripensamento alla copertura delle esigenze finanziarie delle aree protette e una generale regionalizzazione delle aree protette nazionali. Sono questioni, queste, che il disegno di legge n. 119 non affronta minimamente. Ricordo che, nella scorsa legislatura, si è parlato della possibilità dì trasformare gli enti parco in associazioni o in fondazioni e anche di trasformare gli enti parco nazionali in enti regionali, prevedendo i finanziamenti attraverso il federalismo fiscale. Si tratta di problematiche in cui il disegno di legge n. 119 non interviene minimamente. Altro elemento per noi non condivisibile è il fatto che l'articolo 7 del disegno di legge in parola limita ulteriormente i prelievi faunistici e gli eventuali abbattimenti selettivi,

una direzione diametralmente opposta a quella da noi auspicata; meglio allora lasciare che tali questioni siano affrontate direttamente dagli enti parco, nell'ambito dei regolamenti di parco. Si tratta quindi di un'ulteriore centralizzazione, che va nella direzione opposta a quella tracciata dalla Lega Nord. In conclusione, sia per le ragioni esposte, che entrano nel merito del provvedimento, che con la procedura d'urgenza seguirà un esame abbreviato che comprimerà il dibattito generale, sia perché entro fine anno dovrebbe realizzarsi la conferenza, annunciata dal Ministro dell'ambiente, su aree protette, biodiversità

per introdurre eventuali modifiche e arrivare ad un testo che sia concorde con gli

rendersi conto che adottare una procedura d'urgenza non vuol dire fare un lavoro affrettato, ma vuol dire avere la consapevolezza e la determinazione di arrivare in tempi giusti e ragionevoli

BLUNDO *(M5S)*. Presidente, colleghi, il nostro Paese ha molte urgenze: alcune sono vere, perché causate da calamità naturali o derivanti dai bisogni e dalle esigenze dei cittadini;

disconoscendo così le vere urgenze del Paese, che vengono ricordate solo nei salotti televisivi. Mi riferisco, soprattutto, al rilancio dell'occupazione, al ripristino della legalità e dell'etica pubblica come principi cardine della società, alla prevenzione contro i dissesti idrogeologici, alla tutela dell'ambiente, della qualità dell'aria e della salute dei cittadini. È accettabile, tutt'al più, intervenire con urgenza qualora vi sia il bisogno di migliorare qualcosa quando, preso atto in un determinato settore di alcuni vuoti legislativi

Ma in questo disegno di legge sulle aree protette avviene, cari colleghi, esattamente il contrario di quanto appena esposto: le modifiche alla legge quadro n. 394 del 1991 sono nel complesso disomogenee e, come troppo spesso già accaduto in passato, peggiorano sensibilmente la bontà dell'impianto normativo esistente. Il Movimento 5 Stelle non considera intoccabile la legge n. 394 del 1991, ma ritiene che la sua modifica non possa prescindere da una seria ed attenta valutazione sull'applicazione della normativa e sullo stato attuale dei parchi e delle riserve naturali del nostro Paese. Anche il nostro Gruppo ha preparato un disegno di legge in merito, che prevede un'apertura solo nella dimensione ludico-educativa e sportiva, nonché culturale. Prendiamo atto, Presidente, che il metodo seguito in questa legislatura è uguale a quello utilizzato nella precedente. Nonostante non si sia proceduto ad un coinvolgimento ampio di tutti gli attori interessati al rilancio del ruolo dei parchi e delle riserve naturali, passaggio doveroso e necessario a garantire l'efficace conservazione del patrimonio naturale del Paese, si vuole ora agire d'urgenza, limitando persino il confronto dei testi in quest'Aula. Sono molti, poi, gli aspetti del disegno di legge n. 119 che ci lasciano perplessi. Innanzitutto, la distinzione che si vorrebbe introdurre tra attività venatoria e controllo della fauna selvatica, pur con la supervisione dell'ISPRA, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale del Ministero dell'ambiente. Si prevede di fatto, in tal senso, un diretto coinvolgimento dei cacciatori nella gestione della fauna all'interno delle aree naturali protette. La normativa attuale, però, già consente interventi da parte degli enti parco per la gestione dei problemi che alcune specie - essenzialmente il cinghiale - possono determinare se presenti in sovrannumero. La riforma prevista rischia di aprire le porte alla caccia nei parchi, soddisfacendo pertanto interessi che nulla hanno a che fare con la conservazione delle preziose biodiversità nel nostro Paese. Perplessità notevoli destano anche le norme che introducono le *royalty* a favore degli enti gestori, a titolo di compensazione per gli impianti impattanti presenti nei parchi o che si intende realizzare, come il gasdotto SNAM, che ne attraverserebbe molti, tra cui i parchi nazionali della Maiella, dei monti Sibillini e del Gran Sasso e ben 21 fra siti d'interesse comunitario e zone a protezione speciale. queste disposizioni, non valutate a fondo, sono tuttavia atte a determinare pesanti condizionamenti nella gestione delle risorse naturali dei territori protetti, dato che si propone di modificare le procedure di nomina di presidenti e direttori.

Signori, il discorso è articolato e non può essere affrontato con modifiche non organiche alla legge n. 394 del 1991 e, tanto meno, con procedura d'urgenza e rito Per questi motivi, oggi, solennemente voteremo contro questa inopportuna e inaccettabile dichiarazione d'urgenza. altresì un'ampia riflessione, il vostro possibile ripensamento e l'apertura di un vero e leale confronto con tutti gli operatori del settore parchi prima di riavviare, nei tempi e modi opportuni

Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, ho chiesto la parola per intervenire su una situazione che in questo momento preoccupa moltissimo tutti i firmatari dell'interrogazione

da più di due anni dall'inizio del conflitto 100.000 persone hanno perso la vita. Di questi, i bambini uccisi sarebbero ben 7.000, di cui un terzo sotto i dieci anni di età. Inoltre, più di tre milioni di fanciulli sono esposti a rischi di malattie e violenze. secondo i dati, il numero di profughi dall'inizio del conflitto del 2011 in Siria sarebbe di oltre due milioni, rifugiati negli Stati confinanti, e di questi ben un milione sono bambini. Quasi due milioni sono gli allievi della scuola dell'obbligo che hanno abbandonato gli studi nel corso dell'ultimo anno accademico. L'UNICEF si è adoperata nell'assistenza socio‑sanitaria per bambini fuggiti dal conflitto in Libano, Turchia, Giordania, Iraq; ha creato spazi a misura di bambino, dove, oltre all'assistenza tradizionale di tipo materiale (i pasti e il vestiario adeguato) e sanitario, sono presenti spazi gioco, servizi di sostegno psicosociale per i bimbi e gli adolescenti soli e assistenza per il ricongiungimento familiare. Sappiamo di tanti bambini soli provenienti dalla Siria che ogni giorno i banconi sbarcano sulle nostre coste. Dai *media* abbiamo appreso, poi, il 21 agosto in tre ospedali di Damasco, dove erano ricoverati 3.600 pazienti, sono decedute 355 persone e tra queste molti bambini. L'orrore di quelle fotografie è ancora nei nostri occhi. Si è ipotizzato l'uso del gas nervino contro la popolazione e l'indagine terminata il 29 agosto ha dato dei risultati. Sappiamo che il presidente del Consiglio Letta ha ribadito «la più ferma condanna dell'utilizzo di armi chimiche ai danni della popolazione civile siriana quale atto che ripugna la coscienza del popolo italiano e che si configura come crimine contro l'umanità. Tale palese violazione del diritto internazionale è inaccettabile ed i responsabili dovranno essere sottoposti alla giustizia internazionale». Abbiamo sottoscritto diverse Convenzioni, quindi parliamo tantissimo. vorremmo conoscere quali iniziative a livello europeo e internazionale siano in atto da parte del Governo italiano per assicurare da parte delle autorità siriane il rispetto dei diritti civili, politici, economici e sociali stabiliti dalle Convenzioni internazionali sull'infanzia in favore dei fanciulli vittime della guerra. se e quali azioni l'Italia intenda promuovere per potenziare l'intervento umanitario in Siria, salvaguardando la popolazione civile, le donne, gli anziani e in particolare i bambini, al fine di prevenire ulteriori repressioni violente contro gli inermi in Siria. Noi ci siamo distinti e ci distinguiamo anche in questo momento per le azioni umanitarie

un ragazzo perbene che proviene da una famiglia perbene, un'eccellenza della medicina, un urologo di grandi prospettive. Ebbene, nel 2004 Attilio, che oggi avrebbe grosso modo la mia età, è stato trovato morto. Le indagini - che non voglio qualificare e che, per il ruolo che ricopro, non posso fare altro che accettare ma non condividere, perché piene di lacune

2003 venne operato in un ospedale di Marsiglia. Ebbene, nel 2003 Attilio si trovava proprio a Marsiglia.

Signor Presidente, non c'è cosa peggiore che trovarsi da cittadini qualunque a combattere da soli contro la mafia, ed è quello che è successo alla famiglia Manca.

Non può essere messo tutto a tacere così: oggi una mamma e tutta una città

episodi in quasi tutti gli alberghi, furti in 14 strutture turistiche, altri casi sventati casualmente.

non lasciare questi territori in preda a nuove organizzazioni criminali, perché di questo si sta trattando. In altre zone sappiamo che la criminalità organizzata gestisce il territorio; dalle nostre parti, per fortuna, questo non avviene. Vorremmo scongiurare un'ipotesi del genere. Il Ministro della difesa potenzi al massimo la presenza delle forze dell'ordine, perché l'alternativa sarebbe la giustizia fai da te. Dalle nostre parti non si accetta questo stato di cose. *(Applausi

Questi subiscono interferenze nelle decisioni fondamentali, politiche, economiche e militari da parte di organizzazioni mondiali che non dipendono da nessuno Stato. Per le loro attività non rispondono a nessun Governo, non sono sottoposte al controllo di nessun Parlamento e di nessuna istituzione che rappresenti l'interesse collettivo. In poche parole, la struttura politica del mondo sta per essere sconvolta. Le grandi imprese multinazionali non solo attentano agli interessi dei Paesi in via di sviluppo, ma la loro azione incontrollata e dominatrice agisce anche nei Paesi industrializzati in cui hanno sede. La fiducia in noi stessi, che incrementa la nostra fede nei grandi valori dell'umanità, ci dà la certezza che questi valori dovranno prevalere e non potranno essere distrutti».